la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. Vedo con piacere che è ritornato il vice presidente Calderoli, cui do il benvenuto a nome di tutti.

ricorderete che, a seguito della seduta dell'Assemblea dello scorso 3 agosto, la Presidenza fu investita della richiesta di fare luce su presunte espressioni verbali

visionando le immagini a disposizione. Al termine di tale accertamento comunico che non è emerso alcun elemento sindacabile attribuibile alla vice presidente Taverna nel corso

Con questo ritengo pertanto chiuso tale episodio.

Signor Presidente, purtroppo ieri sera siamo stati raggiunti da una pessima notizia: è scomparso Carlo Dell'Aringa, portato via purtroppo da un malore improvviso. Era un nostro collega, uno dei nostri, della nostra comunità del Partito Democratico. Era un docente appassionato ed era soprattutto un uomo gentile. È stato tante cose, ha ricoperto diversi ruoli. Si è formato a Milano, ha studiato scienze politiche all'Università Cattolica, si è poi specializzato all'estero in economia e alla Cattolica ha fatto tutta la sua carriera accademica, diventando giovanissimo ordinario di economia politica e poi fondando negli anni Ottanta un laboratorio, un pensatoio si direbbe oggi, cioè il Centro di ricerche economiche per i problemi del lavoro e dell'industria. Proprio sui problemi del lavoro tanti di noi l'hanno conosciuto

e poi lo ha fatto in Parlamento, quando nel 2013 il Partito Democratico gli chiese di candidarsi in Lombardia, e come Sottosegretario durante il governo Letta. Questi incarichi li ha svolti con il suo stile, con il suo profilo caratteriale. Carlo era una persona che non amava la politica urlata, la politica sguaiata; amava studiare e approfondire, era un politico serio, competente e appassionato. Mite lo definirebbero i più, ma di quella mitezza che non è da scambiare per arrendevolezza, perché era determinato e chi lo ha conosciuto lo può testimoniare. Quando l'ho incontrato nei cinque anni in cui abbiamo lavorato insieme, mi colpiva, nei confronti e nelle discussioni che avevamo, l'eleganza nei modi e nei pensieri; e questo dovrebbe farci pensare, in un periodo come questo in cui lo scontro, spesso sguaiato, come dicevo prima, prevale sul rispetto reciproco. Lui era lontano anni luce da quel tipo di politica. In queste ore vorrei che ai familiari giungesse l'abbraccio dei colleghi del Partito Democratico e non solo, di tutti coloro che l'hanno conosciuto e che hanno fatto con lui un tratto di strada insieme. Un pensiero speciale a te, Carlo. Che il tuo esempio e il tuo stile ci sia di ispirazione nel nostro impegno politico. Ne abbiamo davvero bisogno.

Signor Presidente, colleghi, molti di voi sanno quanto noi ostinatamente alla presentazione di decreti

invece, ci troviamo di fronte a un decreto-legge che in modo molto confusionario, sia nella prima versione e a maggior ragione nelle modifiche introdotte durante il passaggio alla Camera, mette insieme una serie di norme che incidono sui settori più svariati: dalle funzioni fondamentali dei Comuni, all'irrilevanza del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di di riequilibrio, alla proroga dei termini per la conclusione dei lavori della commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni. Esso è inoltre intervenuto pesantemente su alcune materie

fatto sempre rilevare l'incostituzionalità di decreti-legge cosiddetti milleproroghe, che peraltro rappresentano, a nostro avviso, nei fatti, una sorta di fallimento dell'amministrazione

come secondo atto importante del «Governo del cambiamento» onestamente questa è stata davvero una sorpresa. Un'altra sorpresa è stata che, all'interno di questo milleproroghe, si è, in un modo o nell'altro, surrettiziamente, tentato di immettere elementi che forse volevano preludere a interventi di più ampia portata, rinunciando nei fatti, attraverso questi interventi *spot*, a

il decreto stesso e ancor di più, signor Presidente e colleghi, introducono elementi a nostro avviso di palese incostituzionalità. Penso, ad esempio, a quanto è accaduto per quanto riguarda la vicenda dei vaccini. Se il Governo aveva intenzione di modificare le norme sui vaccini, avrebbe dovuto assumersi la responsabilità

sul decreto Lorenzin). Se c'erano questioni da affrontare, certamente bisognava assumersi questa responsabilità politica. Invece abbiamo visto solo confusione, che ha creato problemi nei cittadini, nei genitori, nelle scuole. Al Senato viene presentato e approvato un emendamento con cui si interviene sull'obbligatorietà per quanto riguarda la scuola dell'infanzia;

all'interno di norme che siano chiare e che non mettano, con la loro stessa confusione, a repentaglio la certezza; perché - guardate - in materia sanitaria la certezza del diritto e delle norme è assolutamente necessaria. Arriviamo a un altro intervento: sempre al Senato era stato approvato un emendamento che riguardava la riapertura delle

trattava di uno strumento a disposizione per poter intervenire sulla vicenda dei diplomati magistrali e su altre vicende che riguardano 40.000-50.000 persone, insegnanti che hanno garantito in tutti questi anni la continuità didattica.

all'articolo 13, che è stato oggetto qui al Senato di un intervento anche in questo caso molto confuso, di cui alcuni membri del Governo danno un'interpretazione e altri membri del Governo ne danno un'altra. Sta di fatto che si è intervenuti pesantemente su risorse su cui i Comuni avevano fatto ampio affidamento, anche in questo caso limitando di fatto la facoltà dei

il nuovo Regolamento ci consente di fare un ragionamento un po' più ampio, nel merito dei contenuti e anche nel merito politico, che ci portano a chiedere che il decreto-legge non venga discusso e votato. Sono stati giorni difficili, con una maggioranza tutta tesa a silenziare i toni e la discussione, fino ad arrivare, pur in mancanza di contraddittorio e di interlocuzione, a chiudere ad ogni discorso ed espressione dell'opposizione. Perché questo atteggiamento? Per coprire e far passare in secondo piano le scelte negative contenute nel decreto-legge. Si tratta di scelte negative per le comunità locali, per i cittadini, per le famiglie, famiglie, fatte in molti casi senza neppure esplicitarne il senso e la visione. Forse è troppo chiedere qual è la visione, è troppo chiedere qual è la visione, perché ogni giorno vediamo in campo non uno, ma due Governi, che agitano per aria in modo alternato un contratto, che ad oggi pare un libro dei sogni, che per il momento sta producendo solo lo smantellamento di molte azioni, che agli occhi di tanti sono giuste e di buon senso. Non esito a definirla una sorta di furia ideologica, che anche nel caso di questo sciagurato milleproroghe si manifesta in modo eclatante su due temi, che voglio sottolineare. Innanzitutto l'ambiguità del Governo e della maggioranza sui fondi per le periferie, che si è svelata essere una precisa volontà di togliere i fondi per tanti interventi di grande valore infrastrutturale, sociale urbanistico, di rammendo e di qualificazione proposti da 87 Comuni e 9 Città metropolitane, da Nord a Sud. Ad una formulazione possibilista, il Governo e la maggioranza hanno poi evitato ripetutamente di fornire un'interpretazione chiarificatrice sulla disponibilità dei fondi per i progetti finanziati. Se in questi due giorni, in Commissione, abbiamo usato il tempo a disposizione per evidenziare l'importanza dei fondi per le periferie, era anche per dare tempo al Governo per fare un passo in avanti e chiarire a tutti, al Parlamento e ai sindaci dei Comuni, quale fosse la propria volontà con un ordine del giorno, un semplice ordine del giorno. Lo dico ai colleghi di Lega e 5 Stelle ma anche ai colleghi di Forza Italia, perché non si tratta solo di modi diversi di fare ostruzionismo. Noi siamo qui per consentire un contributo di chiarezza, per migliorare i provvedimenti. Questo è il ruolo dell'opposizione e noi vogliamo farlo fino in fondo perché la presenza dell'opposizione nelle democrazie dà qualità anche all'azione di Governo. Ma qui, ormai, di opposizione mi pare che oltre al Partito Democratico e a LeU ci sia poco altro all'orizzonte, con la Lega che manovra sia il Governo sia l'opposizione di centrodestra. i vaccini, voglio ripetere due cose che siamo riusciti - bontà loro - a dire in Commissione: sono iniziate le scuole e arrivano i fatti. Spostano i bambini immunodepressi dalle classi in funzione della percentuale di vaccinati. Addirittura a Rimini hanno spostato alcuni bambini per ridurre i rischi per il loro papà immunodepresso. Vede, signor Presidente, lo dico a tutti: abbiamo un sistema sanitario che reagisce anche alle vostre scelte sconsiderate perché assume iniziative che vanno a ridurre il rischio.

Sono i medici e i dirigenti scolastici che cercano di ridurre i rischi che voi avete aumentato. Saremmo allora noi a fare ostruzionismo? No! Siete voi che fate ostruzionismo al buon senso, alla scienza e alla salute degli italiani. Vi siete proposti, come cittadini, di essere dalla parte dei cittadini? Con queste scelte siete contro i cittadini. Avete preso i voti dicendo «prima gli italiani»? Con queste scelte siete contro gli italiani. porre una pregiudiziale, oggi, significhi cercare ancora una volta di rendere tutti consapevoli di alcuni temi importanti che in questo decreto milleproroghe vengono trattati in una maniera assolutamente negativa per il nostro Paese. Per questo voteremo a favore della questione pregiudiziale. Ha facoltà di parlare il senatore Pagano per illustrare la questione pregiudiziale QP4.

dagli enti territoriali alla giustizia, dal tema ambientale al settore delle infrastrutture. Sono poi previste proroghe di termini relativi a interventi emergenziali nei territori colpiti dagli eventi sismici, in materia di istruzione e università, di politiche sociali, cultura, sport e nel delicato settore della salute, così come si interviene nuovamente in materia di banche popolari; decreto-legge, è adottato da ormai tutti i Governi, di norma con periodicità annuale, adducendo quale unica giustificazione la necessità di assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'azione delle diverse amministrazioni interessate, ma in realtà serve unicamente a correggere errori, compensare ritardi e mancate decisioni; il continuo e reiterato uso della decretazione d'urgenza si configura, peraltro, come una forma di sbilanciamento e di forzatura degli equilibri dei poteri previsti dall'articolo 70 del dettato Costituzionale, che ha spostato di fatto in capo al Governo ogni potere legislativo ed imposto una compressione delle prerogative delle Camere con buona pace del confronto democratico, diventato quasi del tutto aleatorio; dalla data di insediamento del nuovo Governo, in soli due mesi sono stati presentati ben dieci decreti-legge, nessuno con i requisiti di necessità e urgenza richiesti, non è chiaro quale sia la programmazione politica, nel breve e lungo termine, di questo Governo, che continua a sbandierare un programma ricco di propaganda, ma con pochi - e allarmanti - punti operativi. Non vogliamo credere che il nostro Paese viva in una situazione di emergenza costante; ciò stupisce ancora di più se si pensa che proprio la componente politica dell'attuale Governo, nell'illustrazione della questione pregiudiziale dell'ultimo decreto «milleproroghe», denunciava «l'ennesimo utilizzo di uno strumento, quello appunto della proroga dei termini, che per sua natura già dovrebbe avere un carattere di eccezionalità, ma assume ormai nel nostro Paese un carattere sistematico ed un appuntamento fisso, anno dopo anno, come una prassi ormai consolidata. Il Governo Renzi, che tanto vuole far credere ai cittadini di avere un carattere riformatore, invece nell'utilizzo dell'ennesimo decreto milleproroghe si dimostra il più conservatore dei Governi di sempre, sotto le vesti di giovani governanti che, invece, nascondono le più vecchie strutture di Stato che, per l'ennesima volta, ricorrono al decreto milleproroghe per poter differire i termini di legge completamente disattesi.»; è cambiato il maggioranza di Governo, nei confronti del Governo a guida PD. Dobbiamo registrare che è cambiato il Governo, ma non è cambiato il modo abusato di ricorrere all'utilizzo di questo strumento, e quindi alla violazione della Carta costituzionale. Come veniva sottolineato dalla senatrice De Petris, l'eterogeneità delle materia rappresenta ovviamente per noi il motivo per il quale sosteniamo l'incostituzionalità

l'omogeneità dei contenuti del provvedimento va valutata sia con riferimento alla materia oggetto di disciplina che da un punto di vista teleologico, con riguardo, pertanto, al fine unitario dell'intervento; dall'esame delle singole disposizioni emergono, invece, molteplici finalità, così come interventi su termini fissati dallo stesso Governo con provvedimenti presentati, e approvati in tutta fretta, solo poche settimane prima. È il caso, piuttosto eclatante, dell'articolo 9, che proroga i termini per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e delle eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite. Non serve ricordare che nemmeno due mesi fa, il 19 luglio, questo Parlamento ha approvato in via definitiva il disegno di legge «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche

l'articolo 6, come modificato in sede di esame dal Senato, che ha previsto la possibilità per gli insegnanti abilitati entro l'anno 2017-2018 e per coloro che sono in possesso del diploma magistrale conseguito entro il 2001-2002 o di un diploma che dà accesso al profilo di insegnante tecnico-pratico, di inserirsi una fascia aggiuntiva delle GAE. Voglio ricordare le promesse fatte in campagna elettorale al mondo della scuola: questi insegnanti sono stati prima illusi e poi delusi in maniera clamorosa, vista la confusione pazzesca che c'è stata qui in Aula. Noi condividiamo l'emendamento della senatrice De Petris, che peraltro, in questa materia, viene a contraddire, secondo le intenzioni del Governo, ciò che invece è previsto dal decreto dignità. Non meno gravi sono le previsioni che riguardano le Province italiane: la legge Delrio è stata un esempio di psichiatria politica e di psichiatria legislativa. Oggi si passa alla legislazione creativa: le elezioni che vengono indette al 31 ottobre, noi ci troveremo a votare in molte Province soltanto per il Presidente, mentre in molte altre i consigli provinciali verranno sciolti in maniera anticipata rispetto alla loro scadenza naturale per una fretta inspiegabile. Noi inoltriamo nuovamente l'invito alla maggioranza di Governo ad approvare una legge che ridia voce al popolo e faccia in modo che i Presidenti delle Province e i consigli provinciali tornino a essere scelti dai cittadini. Quello che stiamo vedendo nelle Province aggiunge confusione alla grande confusione che è stata creata dalla cosiddetta legge Delrio, ribattezzata "delirio". Anche le norme in materia di proroga di banche popolari e le norme in materia di proroga degli obblighi vaccinali rappresentano un motivo forte per il quale siamo contrari a questo decreto *omnibus* e per il quale chiediamo all'Assemblea del Senato di deliberare di non procedere all'esame del disegno di legge.

Signor Presidente, la ringrazio per avermi concesso la parola. Non è la prima volta che il Gruppo di Forza Italia presenta una questione pregiudiziale al milleproroghe. È già accaduto in prima lettura, ma è evidente che la questione non è di lana caprina. Non è un problema, quello della pregiudiziale, che può essere taciuto, quando si tratta in modo chiaro di un caso di abuso di decretazione d'urgenza; un fatto evidente che reca un danno all'attività legislativa del Parlamento. Nel corso della prima lettura erano già chiare ed evidenti tutte le disposizioni legislative contenute all'interno di questo provvedimento definito milleproroghe, appare divenuto ormai una consuetudine per il Parlamento. È un aspetto che noi dobbiamo rilevare come un fatto negativo:

come l'attuale maggioranza afferma, che si vogliono cambiare tutte le cattive abitudini del passato, allora la prima cattiva abitudine che c'è stata negli anni e nelle legislature del passato è proprio quella di far ricorso in modo

della sua emanazione con cadenza sistematica, in quanto ormai divenuta una prassi consolidata del Parlamento, costituisce evidentemente un fortissimo disincentivo per la pubblica amministrazione che invece di adempiere ai propri doveri, sa già, prima ancora che i termini scadano, che tanto arriva il milleproroghe di turno ed è questo il modo per poter superare le scadenze che che intervengono e che devono essere invece assolutamente rispettate per una buona amministrazione e per un buon Governo. Capite bene che tutto questo non può più proseguire;

vicepresidente della 1a Commissione, ha fatto rilevare in Commissione come, in effetti, in prima lettura alcune modifiche sono state richieste e non approvate, mentre alla Camera dei Deputati l'attuale maggioranza e il Governo italiano abbiano posto alcune modifiche, anche significative, che certamente fanno intuire un fondo di incertezza rispetto al percorso che la maggioranza dovrebbe dare all'Italia.

che prende continuamente sbandate, una volta sterza a sinistra e una a destra, perdendo il controllo dell'auto; dove andiamo a sbattere? Non è più possibile pensare a tutto questo. Pertanto, dico francamente che le modifiche intervenute in prima lettura alla Camera dei deputati, quindi nel secondo ramo del Parlamento, non ci piacciono; quella che in particolare non ci piace riguarda la nota questione dei vaccini. È giusto ricordare come il Gruppo Forza Italia, già in prima lettura al Senato, ne abbia fatto una battaglia di civiltà, che non vuol dire soltanto seguire in modo pedissequo e comunque senza osservazione il mondo della scienza medica; significa semplicemente essere moderni, vicini al Paese, far in modo che esso guardi al futuro con speranza e che miri soprattutto

alla Camera dei deputati, quando sembrò che la maggioranza stesse modificando il proprio approccio a questo provvedimento, di fatto poi ha deluso perché, in realtà, è stata solo inserita una proroga, fino al 10 marzo 2019, del termine per consentire la possibilità di presentare l'autocertificazione. In sostanza, è un modo per non assumere una posizione chiara,

che a noi interessa, del bando delle periferie: un bando annunciato, per il quale alcune amministrazioni locali (non poche: 87 Comuni capoluogo, 9 Città metropolitane 1.625 interventi che riguardano un totale di 326 Comuni) avevano già avanzato delle iniziative affinché si potesse venire incontro

cara collega Bernini, ha ripresentato un emendamento, nella speranza che ce lo facciano votare e possa essere approvato. Ma concludo con la questione degli edifici scolastici. Anche sugli edifici scolastici il provvedimento modificativo (e l'ho detto anche in Commissione al Sottosegretario, che amabilmente mi ha risposto) è insufficiente rispetto all'assoluta necessità di far sì che tutti gli edifici scolastici possano essere

Colleghi parlamentari, il provvedimento, per le ragioni di merito e di forma, e innanzitutto per le ragioni di diritto, è viziato sia dal punto di vista della legittimità costituzionale, sia perché ha un contenuto disomogeneo (in quanto si preoccupa di troppi argomenti in modo scollegato l'uno dall'altro), sia perché privo dei requisiti straordinari di necessità e di urgenza. *(Applausi

Sono presenti in tribuna Giovanni e Ilaria Tesse, fratello e sorella, di quattordici e dodici anni, giovanissimi campioni italiani di danze latine 2017 nell'ambito della Federazione italiana di danza sportiva.

Presidente, colleghi, noi siamo fortemente contrari a questo provvedimento, perché pensiamo che esso contenga tre violenze e due gravi omissioni. Le violenze che questo provvedimento contiene sono dirette contro il diritto alla salute dei bambini e delle famiglie di questo Paese, contro il diritto all'istruzione e contro i Comuni italiani. Le due gravi omissioni riguardano ciò che si è deciso di non fare per rafforzare gli aiuti alle popolazioni colpite dal terremoto e per rafforzare e accelerare i supporti decisi in favore dei risparmiatori colpiti dalle truffe delle banche. Noi in questi giorni abbiamo cercato, in 1a Commissione affari costituzionali, dove io sono Capogruppo del Partito Democratico, di far aprire gli occhi alla maggioranza e al Governo sui limiti evidenti di questo provvedimento. Abbiamo cercato di ottenere miglioramenti (è dovere dell'opposizione farlo), abbiamo prospettato argomenti e abbiamo avanzato istanze di modifica. Non ci è stato possibile ottenere alcuna risposta costruttiva: sordità alle nostre richieste e mutismo, che si è trasformato nella decisione del Governo e della maggioranza, molto grave, di non alimentare il dibattito in Commissione, di non partecipare al confronto che noi proponevamo e di segnare quindi una pagina non positiva della storia della 1a Commissione e di questo Parlamento. Noi abbiamo fatto molti interventi, tutti di merito, tutti attenti alla sostanza, portando esempi concreti. Abbiamo fatto capire che la decisione sul bando periferie significherà asili che non saranno fatti, scuole che non saranno ristrutturate o costruite, strade che non saranno realizzate; significherà città più insicure; significherà maggiore incertezza per i Comuni italiani. E, quando noi infliggiamo ai Comuni maggiore incertezza, dobbiamo sapere che una fonte rilevantissima

E che dire di quanto è stato fatto sui vaccini: voltafaccia, piroette, continue dichiarazioni, che hanno prima confuso le idee a gran parte dell'opinione pubblica e poi hanno reso chiaro, con la decisione finale, che questa maggioranza e questo Governo sono contrari al diritto delle famiglie e dei bambini di veder salvaguardata la propria salute. E lo sono in maniera più grave se teniamo presente il fatto che la comunità scientifica, il mondo della cultura e il mondo della scuola hanno fatto presente quanto non si dovesse percorrere la strada che si è deciso di percorrere. Pertanto, credo che le ragioni di contenuto che ho appena illustrato e le ragioni di metodo che si è deciso di seguire nella discussione di questo provvedimento rendano necessari la continuazione della battaglia dell'opposizione durante la discussione plenaria in Aula e anche, successivamente al voto sul provvedimento, nel Paese, perché ci sono cose sulle quali siamo consapevoli di poter contare su un appoggio che va ben oltre la cerchia dei parlamentari che compongono i Gruppi di minoranza in questo Parlamento. Ci possiamo collegare ai mondi che ho citato prima, quello della scuola, quello dei sindaci, quello della cultura, a tutte le persone che ritengono si debba far prevalere la ragionevolezza sull'ideologia e su un approccio demagogico ai problemi. Abbiamo assistito, durante i lavori svolti in Commissione su questo provvedimento, situazioni molto spiacevoli: ci è stato dato pochissimo tempo per preparare i nostri emendamenti, con una forzatura che tutti abbiamo trovato assolutamente infondata e non ragionevole. Si è deciso, in Commissione bilancio, di adottare un ricorso sistematico, improprio e - non esito a dirlo - abusivo all'articolo 81 della Costituzione per far decadere in massa emendamenti ed impedire che su di essi ci fosse una riflessione sufficientemente approfondita fino a costringere i Gruppi di opposizione ad uscire dalla Commissione, così come abbiamo dovuto fare noi quando c'è stata la forzatura in 1a Commissione sugli emendamenti. la decisione del Presidente della 1a Commissione di troncare inopinatamente il dibattito in Commissione prima che si fosse esaurita la discussione, quando questo decreto-legge ha per scadenza la prossima domenica e, se si fosse voluto, soprattutto alla luce di quanto il nuovo Regolamento del Senato consente alla maggioranza in termini di velocizzazione dei lavori in Assemblea, si sarebbe potuto utilizzare la giornata di oggi e quella di domani, facendo arrivare il provvedimento in tempo utile per l'approvazione prima della sua scadenza. Invece no: si è applicata una sorta di mannaia ai lavori della Commissione; si è voluto strozzare il dibattito; si è voluta dare un'ulteriore prova di protervia e di arroganza. Noi a tutto questo ci opponiamo, non soltanto ai contenuti del provvedimento. Invitiamo tutti a riflettere su come le forzature siano sempre sbagliate e su come, quando non sono necessarie, diventino ancora più sbagliate. Voglio affrontare un ultimo punto. Con il bando periferie non si è creata soltanto incertezza sulle decisioni di investimento dei Comuni, ma si è infranto, a mio avviso, un principio fondamentale dell'ordinamento di qualsiasi democrazia ben funzionante: la continuità dello Stato pur nel mutare e nella discontinuità delle maggioranze. Non si rimettono in discussione fondi già assegnati; non si rimettono in discussione decisioni già prese per seguire un capriccio spartitorio o di altro tipo. Lo Stato non cambia le carte in tavola; tavola; se lo Stato cambia le carte in tavola, perde autorevolezza e credibilità, e trasmette ai livelli istituzionali inferiori un segnale di confusione e di mancanza di certezza del diritto che può far soltanto male alle imprese e alle famiglie di questo Paese.

della continuità e del buon esito di questa legislatura. Farò dei riferimenti molto specifici e puntuali, partendo ovviamente

abbiamo cominciato i lavori nel pomeriggio di lunedì, signor Presidente, ed in Commissione è stato deciso di fissare i termini per la presentazione degli emendamenti: in maniera incomprensibile, anche da un punto di vista dell'utilità della maggioranza e di capacità di lavoro degli uffici, è stato volontariamente impedito al Partito Democratico di avere tempi sufficienti per affrontare le tante le tante modifiche intervenute alla Camera, quando si è voluto forzatamente fissare un termine molto breve la sera stessa. Dopo c'era la notte e gli uffici non avrebbero lavorato; noi chiedevamo quindi di poter lavorare tutta la notte per preparare i nostri emendamenti. comportamento sia lesivo anche, e forse soprattutto, perché non vi era nessuna ragione pratica né politica per addivenire a questa decisione; c'era solo la volontà di impedire al nostro Gruppo, ai nostri uffici, di lavorare con sufficiente tempo alla preparazione degli emendamenti e degli ordini del giorno.

specifico e ci comunicò di aver provveduto a parlare con il Ministro competente, il ministro Tria, e con il Presidente della Commissione, affinché non si ripetessero quelle situazioni

c'è stato un vaglio preventivo, se c'è stata una verifica con la Presidenza del Senato. Qual è la situazione? La terza situazione che giudichiamo preoccupante per l'andamento della vita democratica dell'Assemblea per la seconda volta, su un provvedimento importante voluto dal Governo, arriviamo in Assemblea senza relatore. Comprendiamo che quella sia una *extrema ratio:* ratio:* quando si sono esauriti i tempi, quando la Presidenza ha portato avanti i lavori fino al punto di non ritorno, quando ciò diventa evidente, per esempio nello specifico di un decreto-legge, si può arrivare alla conseguenza logica di approdare in Assemblea senza il relatore, perché altrimenti il provvedimento scadrebbe. Ma non c'erano queste condizioni. Signor Presidente, non c'erano affatto. C'era la possibilità di lavorare in Commissione rispettando il nuovo Regolamento, che prevede proprio in quel luogo l'approfondimento, il dibattito e il confronto. Si è volutamente negato

C'era tempo per svolgere il lavoro nelle Commissioni, anche dando spazio alle opposizioni, incluso un atteggiamento di ostruzionismo che ci imputano, ma questo è legittimo. Si poteva venire in Aula senza il relatore solo nel momento in cui tutti i termini possibili erano esauriti. Invece, si è scelto per la seconda volta - già lo abbiamo denunciato - di impedire alle opposizioni di confrontarsi su questioni rilevanti per il Paese

dei lavori stessi in quella sede, solo come segnale da dare alla Presidenza perché affronti questi temi. Noi abbiamo il diritto di essere tutelati rispetto a questo atteggiamento che va oltre le regole della democrazia e oltre il tollerabile.

Noi pensavamo che questo intervento avrebbe riportato il lavoro della Commissione bilancio a un corretto utilizzo.

dell'articolo 81, con la scusa che non erano arrivate le relazioni tecniche. Noi stiamo per entrare nella sessione di bilancio ed è evidente

che vogliono presentare un emendamento sono messi a repentaglio. Signor Presidente, le chiedo, ancora una volta, formalmente, nello stigmatizzare

Per quanto riguarda la questione del provvedimento che arriva in Assemblea senza il relatore, ritengo - ho sempre ritenuto

non solo per avere la possibilità di stare nei tempi, perché il provvedimento era venuto in Assemblea, ma anche per evitare di arrivare a una discussione approfondita in Commissione. È stato abusato in passato e noi ci siamo sempre opposti. Non vorrei che, anche all'inizio di questa legislatura

emendamenti. Credo che dovremmo ricordarlo tutti in quest'Aula, tanto più perché molti lo hanno già subito pesantemente in passato.

per il Gruppo Forza Italia, devo stigmatizzare, replicando le osservazioni che sono già state fatte anche in corso della Conferenza dei Capigruppo, quello che, nella sostanza, hanno anticipato i colleghi che mi hanno preceduto.

presuntivamente assente relazione tecnica, è una prassi che non possiamo accettare. Lo abbiamo detto molto civilmente, signor Presidente, e lei ce ne deve dare atto. deve dare atto. In occasione di due Conferenze dei Capigruppo abbiamo detto che, essendo cambiato il Regolamento del Senato, tutto ciò che da adesso in poi viene praticato nelle Commissioni, come in Aula - ma soprattutto nelle Commissioni, dove si svolgerà la parte più significativa dell'*iter* di formazione della legge - rischia di assumere natura di precedente. Noi non possiamo più accettare queste male pratiche. Per quanto ci riguarda, per qualsiasi provvedimento, dal decreto dignità fino al decreto milleproroghe che stiamo affrontando ora, abbiamo assunto un ruolo - questo ce lo riconoscono tutti i colleghi, di maggioranza e di minoranza di opposizione assolutamente responsabile, sui contenuti, non isterica, non strumentale, ostruzionistica quanto è opportuno e necessario per il sostegno delle nostre posizioni politiche, nelle quali crediamo in modo particolare, soprattutto a fronte di temi, caldissimi, che sono stati affrontati

che abbiamo concordato in Conferenza dei Capigruppo, nella discussione generale e nella discussione dei singoli emendamenti, se il provvedimento seguirà in Assemblea il suo *iter* normale. Tutto ciò premesso, signor Presidente e colleghi, non possiamo però accettare che in 5ª Commissione i nostri emendamenti, civilmente elaborati e discussi, vengano votati a botte di cento alla volta.

Colleghi, signor Presidente, tutto questo ha ancora una volta uno scopo costruttivo: non permetteremo che passi questa prassi

anche nei tempi più cupi di queste Aule parlamentari, siano rispettati ora, in modo particolare ora, in un momento in cui purtroppo la funzione del Parlamento rischia di essere fortemente indebolita. In ordine alle questioni che sono state poste, la Presidenza si riserva di effettuare gli opportuni accertamenti. il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, oggi all'esame dell'Assemblea, è stato approvato con modificazioni dal Senato il 6 agosto e ulteriormente modificato, in seconda lettura, dalla Camera dei deputati, che ne ha concluso l'esame il 14 settembre. In quella stessa data il disegno di legge è stato quindi trasmesso nuovamente al Senato per l'esame in terza lettura e assegnato in sede referente alla Commissione affari costituzionali. La Commissione ne ha iniziato la trattazione alle ore 18 di lunedì 17 settembre, con la relazione introduttiva e la discussione generale. Anche in vista dell'imminente scadenza dei termini costituzionalmente previsti per la conversione in legge del decreto - il 23 settembre - e per assicurare tempi congrui di discussione e di esame, il termine per la presentazione di emendamenti è stato fissato alle ore 23 dello stesso giorno. Alla scadenza risultavano presenti 84 ordini del giorno e 414 emendamenti. Nella seduta pomeridiana di ieri, martedì 18 settembre, ha avuto inizio l'esame degli emendamenti, con l'illustrazione dei relativi proponenti; fase che è proseguita, come da calendario, nella seduta notturna di ieri e nella seduta antimeridiana di oggi. Alle ore 11 di questa mattina si è preso atto dell'impossibilità di concludere l'esame in tempo utile per l'inizio della trattazione in Assemblea, previsto in base alle determinazioni della Conferenza dei Capigruppo per le ore 18 di oggi. Alle ore 11 di oggi, infatti, ancora era in corso l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 9. Risultava pertanto evidente che, nel tempo che residuava prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, la Commissione non avrebbe potuto completare l'illustrazione di tutti gli emendamenti e, conseguentemente, procedere alle relative votazioni e al conferimento del mandato al relatore. Dalla sintetica ricognizione dell'esame in Commissione ritengo di poter affermare che, per quanto serrati in ragione degli imminenti termini per la conversione del decreto-legge, gli spazi di discussione non siano stati compressi. Nelle circa dieci ore di attività della Commissione si sono svolti circa 80 interventi, in gran parte dedicati alle illustrazioni delle proposte emendative. Peraltro, ricordo che la Commissione ha accolto all'unanimità la richiesta avanzata dal Gruppo Partito Democratico all'inizio dell'*iter* affinché l'esame fosse assistito

Onorevoli colleghi, in relazione a quanto riferito dal senatore Borghesi, il disegno di legge n. 717-B, non essendosi concluso l'esame in Commissione, sarà discusso nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati senza relazione, ai sensi dell'articolo 44, comma 3, del Regolamento. Dichiaro aperta la discussione generale. È iscritto a parlare il senatore Causin. Ne ha facoltà. il decreto milleproroghe ha un *focus* molto particolare che tradisce l'identità della maggioranza.

per cui circa 90 città, che avevano vinto regolarmente il bando periferie, si sono viste escluse da un rapporto contrattuale con lo Stato che avevano ottenuto attraverso la partecipazione al bando.

Ci sono due elementi di gravità. In primo luogo, quello che avete compiuto con il milleproroghe è una violazione di un accordo contrattuale tra lo Stato e le città. Quando voi, come maggioranza, rappresentate questo Paese, rappresentate lo Stato. Oltre 90 città avevano già firmato degli accordi, come ha ricordato il collega Pagano. Hanno sottoscritto degli impegni e, a volte, hanno addirittura iniziato a spendere i soldi per riqualificare le aree periferiche degradate. Ma ciò che è più grave che è che il Governo è venuto meno non soltanto a un impegno con le amministrazioni, ma anche a un impegno con milioni di cittadini che vivono in aree degradate del Paese, collocate nelle più grandi aree urbane,

disagio, nel degrado di quelle periferie. E voi state tradendo quei cittadini, quegli elettori negando il finanziamento al bando periferie. lo avete fatto in modo - ripeto - consapevole, in modo determinato; lo avete fatto perché sapete che le finanze dello Stato non consentono in alcun modo di fare la legge di stabilità che avete in mente e lo avete fatto perché volete mantenere delle promesse da mariuoli, promesse da mariuoli, promesse pericolose come - ad esempio - il reddito di cittadinanza, i famosi 780 euro che volete dare alle persone che non lavorano.

a persone che vivono in un Paese dove i servizi di collocamento non funzionano; dove non esistono una formazione professionale e un'economia in grado di assorbire le capacità occupazionali di persone che magari, Voi pensate di poter dare, attraverso quanto previsto nel milleproroghe, attraverso i pochi quattrini che siete riusciti a racimolare,

ai luoghi che sono il volano dell'economia e permettono la tenuta della comunità, la possibilità di investire nella riqualificazione, nell'economia e nella coesione sociale, colpendo associazioni che in questo momento stanno svolgendo compiti e ruoli al posto dello Stato. Questa è una scelta politica consapevole, una scelta politica sbagliata, che, soprattutto, vi si ritorcerà contro.

Il Comune di Bolzano è coinvolto con i 18 milioni che si è aggiudicato per il progetto di recupero dell'areale - in pieno centro - di via Alto Adige. Anche i nostri sindaci hanno duramente protestato contro questa decisione unilaterale del Governo, e spero davvero come promesso dal presidente Conte al presidente dell'ANCI Antonio Decaro - che si trovi quanto prima una soluzione. Bolzano, come Trento, come tutte le altre città interessate, ha bisogno di quelle risorse. Si tratta di finanziamenti già stanziati, bollinati dalla Ragioneria generale dello Stato, che i Comuni stavano cominciando a spendere. Se vi è una necessità di reperire risorse, non è questa la strada giusta, perché parliamo in tal caso di risorse che vanno a diretto e immediato vantaggio dei cittadini. Per questo fatichiamo a comprendere il muro che il Governo ha alzato alla Camera, dopo l'errore che è stato compiuto qui in Senato. È la nota negativa di un provvedimento che ha dei lati anche positivi. Positiva è anzitutto la decisione di prorogare i termini per l'adesione dei gruppi nella riforma delle BCC. In prima lettura, con un nostro emendamento, avevamo chiesto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 La solidarietà per garantire la stabilità del sistema è importante, ma non può arrivare a compromettere la libertà di iniziativa garantita dalla Costituzione e quei principi mutualistici e di connessione col territorio, che costituiscono la ragione sociale del credito cooperativo. Per questo il nostro auspicio è che questo tempo che il Governo si è voluto concedere serva per una riflessione più puntale, attraverso il coinvolgimento e il confronto serrato con i soggetti interessati. Il sistema bancario merita grande attenzione, soprattutto adesso che per le famiglie e le imprese si potrebbe aprire una pagina nuova sul costo del denaro per via della conclusione del *quantitative easing*. Apprezziamo l'atteggiamento prudenziale dell'1,6 per cento, soprattutto in virtù di quello che sta succedendo a livello internazionale e dei dati sulla produzione industriale. L'Italia avrà bisogno di politiche che diano ulteriore slancio alla ripresa; politiche che sappiano conciliare il livello macro con quello micro degli artigiani, dei professionisti, delle piccole imprese. In questo senso, gioca un ruolo fondamentale la semplificazione burocratica che, per i piccoli, assume i contorni di una tassa occulta. Andavano in questa direzione altri emendamenti che avevamo presentato in prima lettura: quelli per il settore agricolo, per prorogare l'entrata in vigore della tracciabilità dei pagamenti, con l'obiettivo di consentire ad ABI e Poste Italiane di sviluppare iniziative volte a ridurne proprio l'impatto burocratico; oppure quello con cui chiedevamo di prorogare di ulteriori sei mesi la scadenza per i nuovi adempimenti delle strutture alberghiere, con il mero scopo di evitare agli albergatori lavori di adeguamento nel pieno della stagione turistica, ossia il giugno del prossimo anno. non è stato possibile in Commissione avviare un confronto adeguato su questi temi. Ne prendiamo atto e auspichiamo che in futuro ci sia una maggiore possibilità di dialogo e confronto, a partire da questioni che non hanno alcuna matrice ideologica se non quella del puro buonsenso. Come abbiamo detto in prima lettura, noi riconosciamo al Governo la possibilità di un provvedimento che serve per approfondire le questioni che reputa più importanti. Ci convince meno quando un proroga-termini quando un proroga-termini perde questa sua funzione originaria e si tramuta in uno strumento per prendere iniziative di cui si fatica a comprenderne la *ratio* e lo spirito d'indirizzo. Il nostro augurio è che la confusione e le retromarce che hanno caratterizzato alcuni momenti dell'esame del provvedimento possano chiudersi qui. Ci attende presto la prima legge di bilancio della nuova legislatura, il primo vero banco di prova di questo Esecutivo. Noi ci confronteremo nel merito - come abbiamo sempre detto - e speriamo di farlo su una legge che trovi il doveroso punto d'equilibrio tra ordine nei conti e impulso alla crescita.

mentre a oggi rimangono irrisolte le questioni sostanziali, relative agli interventi che devono essere fatti. Non c'è ancora - voglio ricordarlo - un Commissario

Questa estate, tra una notizia e un'altra, ho appreso che sia il ministro Di Maio, sia successivamente - se la memoria non mi inganna - il *premier* Conte si sono recati a Ischia e hanno rassicurato il Presidente della Regione e

alla vicenda di Genova - la soluzione anche di alcune questioni relative al terremoto di Ischia. Stando ai fatti,

Noi l'abbiamo sperato perché, del resto, in prima lettura alla Camera dei cambiamenti sono stati fatti. Gli emendamenti sono stati tutti quanti bocciati ed erano emendamenti - come sappiamo - suggeriti dai sindaci, da una parte,

Capite che in queste condizioni, con tutto l'affetto che possiamo avere nei confronti di chi cerca di operare nel bene dello Stato, votare siffatte misure ci è risultato un po' complicato.

la fretta ci ritroviamo ancora una volta in Senato a parlare del milleproroghe.

porti un reale vantaggio ai cittadini italiani e dia un segno di consapevolezza del nuovo Parlamento agli amministratori locali, che sono la prima interfaccia dei nostri cittadini, coloro che sono in prima linea rispetto alle problematiche del quotidiano e a quello che il Paese reale chiede ogni giorno a tutti quanti noi. Purtroppo questa attesa è stata clamorosamente smentita, perché c'è stata una sostanziale questione di fiducia invisibile, come io la definisco. Già nella prima lettura gli spazi per il confronto sono stati assolutamente compressi; non c'è stata la volontà politica di dialogare e di confrontarsi per apportare dei miglioramenti, come era in animo di fare Fratelli d'Italia, una forza politica che ama definirsi di opposizione patriottica, nell'interesse della nostra Nazione. quella fretta ha finito per tradire anche la maggioranza, costretta poi a porre la fiducia alla Camera dei deputati e a tornare qui non senza qualche imbarazzo, così come è avvenuto per ciò che riguarda il mondo dei precari della scuola. Nei mesi di campagna elettorale si sono sprecate le promesse e gli impegni nei confronti delle migliaia di persone che, legittimamente, da anni aspettano una risposta chiara, precisa e - secondo noi - la tutela di un loro diritto di lavoratori.

prevedeva di mettere fuori dal mondo della scuola persone con tanti anni di insegnamento, come nel caso dei diplomati magistrali, è sopraggiunta la politica del reale di quello che si autodefinisce Governo del cambiamento. Anche la confusione che si è generata su alcuni emendamenti oggi ci riporta qui a ridiscutere quello che già ci siamo detti nella prima settimana di agosto. Quello del mondo della scuola, però, è soltanto uno degli aspetti sui quali si poteva e si doveva intervenire in maniera diversa. E lo ripeterò fino alla noia, quello che c'è nell'animo di tanti colleghi, o almeno di quelli che, come me, hanno avuto l'onore e l'onere di essere amministratori delle Province. Noi abbiamo, per colpa della legge Delrio, un livello istituzionale fantasma in Italia. Oggi le Province sono veramente un ente inutile. Non lo erano ieri. noi auspichiamo - e lo avevamo fatto già attraverso la presentazione di emendamenti, che riproponiamo con minore fiducia, purtroppo, in base a quello che si percepisce si metta al centro la questione delle elezioni. Oggi le elezioni per le Province sono veramente poco significative. Si tratta di trovare eroi che vadano a rappresentare un livello istituzionale completamente svuotato della possibilità sostanziale di dare risposte ai territori. Sarebbe stato - e da noi continua a esserlo attraverso la presentazione di un ordine del giorno - un impegno da parte del Governo per tornare all'elezione diretta, diretta, per dare dignità a quel livello istituzionale; un impegno che deve essere immediato, quello sì emergenziale, per dare risposte, in termini di intervento, a migliaia di chilometri di strade provinciali e a scuole medie superiori abbandonate a se stesse. Da anni non ci sono interventi di manutenzione né ordinaria né straordinaria. Non è accettabile che esista un livello istituzionale con funzioni ben precise che, al di là della capacità politica amministrativa dei suoi rappresentanti, non sia nella condizione di operare. Noi abbiamo la responsabilità della sicurezza dei cittadini; abbiamo la responsabilità della sicurezza di migliaia di alunni. E ricordo che da poco è iniziato l'anno scolastico con problemi ovunque sul territorio nazionale. Se non vogliamo essere compartecipi di un errore e di tragedie che non ci auguriamo, dobbiamo avere piena cognizione che deve essere messa mano immediatamente a questo problema. Facciamolo insieme. Sono convinto che vi sia una sensibilità trasversale alle parti politiche, perché ogni giorno tutti noi riceviamo il grido d'allarme dei nostri amministratori locali. E lo stesso grido d'allarme ci viene sulla questione dei fondi per le periferie, una questione assolutamente esiziale per la riqualificazione urbana e per fare in modo che, all'interno della stessa realtà comunale, non ci siano cittadini di serie A e cittadini di serie B. Inoltre, finalizzare queste ingenti risorse significa dare una risposta in termini di riapertura dei cantieri, di rilancio dello sviluppo e di occupazione. Il nostro auspicio è che ci sia ancora spazio per inserire questo confronto. Se la maggioranza lo ritiene, io credo che sia possibile. Signor Presidente, da medico vorrei richiamare ancora una volta l'attenzione di quest'Aula sulla grave responsabilità di chi in questo momento sceglie sceglie di non assicurare con certezza un'adeguata copertura vaccinale ai nostri bambini. Su questo tema negli ultimi anni vi è stata un'ondata di irrazionalità, per cui pochi (veri o presunti) di problemi gravi legati a vaccini sono stati amplificati, creando dubbi e paure. Sono rimbalzate sui *social network fake news* su questo argomento ed è il momento, ora, di recuperare un atteggiamento e un comportamento razionale. I vaccini sono sicuri, e lo sappiamo perché ce lo dice la scienza. sicuri non nel senso che complicanze rare, ma anche gravi, non siano mai possibili. Le complicanze sono possibili, ma la sicurezza deriva dal fatto che le complicanze gravi sono molto rare, a fronte dei grandi benefici dimostrati in termini di riduzione della mortalità e di prevenzione di malattie gravi, invalidanti e potenzialmente mortali. Sicurezza: cosa significa sicurezza? Non significa l'impossibilità di effetti negativi, che corrisponderebbe a un altro pensiero irrazionale, perché tutte o quasi tutte le azioni umane comportano un certo rischio. Saliamo in macchina senza farci problemi, ma gli incidenti ci sono. Anche se camminiamo, prima o poi qualcuno di noi inciamperà. Mangiando, può sempre essere che a qualcuno vada un boccone di traverso. Quindi, è un atteggiamento irrazionale pretendere che sia garantita la sicurezza in termini assoluti. È necessario che la politica recuperi la razionalità e fondi le proprie decisioni sulle evidenze scientifiche migliori che abbiamo disponibili in questo momento; ed esse, a favore delle vaccinazioni, sono solidissime. Vorrei ricordare ancora una volta in quest'Aula alcuni dati, per far nuovamente presente la portata e la rilevanza dell'argomento. Parliamo del morbillo:

di grandezza di un caso su un milione per effetti importanti gravi legati alla vaccinazione. La stessa cosa si può dire La pertosse nei bambini molto piccoli ha una mortalità che si aggira su qualche unità per cento casi di pertosse; arriva invece a causare qualche problema importante in pochi casi su un milione di vaccinati. I vaccini sono farmaci, ovviamente, e come farmaci possono avere effetti collaterali, che però sono di gran lunga inferiori ai farmaci che noi comunemente assumiamo; sono di gran lunga inferiori ad alcuni alimenti: le arachidi che nessuno si è mai sognato di scoraggiare - causano con una certa frequenza reazioni allergiche anche molto gravi e potenzialmente mortali. Quindi è necessario un recupero di razionalità. Oltre alla protezione individuale, Oltre alla protezione individuale, sui vaccini è importante l'immunità di gregge, cioè l'immunità diffusa nella popolazione, garantita da una copertura vaccinale molto elevata, non serve solo a proteggere chi non può vaccinarsi (si è tanto parlato dei bambini immunodepressi), ma serve a proteggere tutta la popolazione, perché, in caso di epidemia, un numero considerevole di casi si verifica nei vaccinati.

decidere, è interesse dell'intera popolazione. Anche per noi sarebbe auspicabile lavorare sulla informazione completa e adeguata, lavorare sulla condivisione, lavorare sulla consapevolezza delle persone. Però quanto è avvenuto, con l'amplificazione di notizie false, il dibattito che c'è stato negli ultimi mesi, il fatto stesso che ci siano dei rinvii dell'obbligo vaccinale, il fatto che questo obbligo diventi «forse» un obbligo e addirittura si senta parlare di obbligo cosiddetto flessibile, flessibile, genera confusione e disorientamento nelle famiglie, tanto che accade frequentemente che genitori, che in precedenza non avrebbero avuto alcun dubbio o problema a vaccinare i propri bambini, adesso si pongono dei dubbi, sono perplessi e non sanno cosa fare. Tutto questo va contro gli obiettivi che si dichiara invece di voler perseguire riguardo a condivisione e consapevolezza.

Signor Presidente, non voglio rinunciare ad intervenire, nonostante sappiamo tutti che il tema che riguarda le Province contenuto nel milleproroghe non darà soddisfazione alla richiesta di tanti amministratori e di tanti sindaci che chiedono di essere tutelati, di avere dignità, di avere un percorso attuabile per le loro istanze. Questo milleproroghe, purtroppo, si conferma una norma che non ha né capo né coda. Che poi sia proroga o anticipo non si capisce bene perché,

ma la risposta non poteva essere quella di rendere impensabile qualsiasi possibilità di dignità delle Province e di azione, facendo in modo che i migliori tecnici scappassero, che non ci fossero le risorse sufficienti, come ho sentito da altri colleghi. Le competenze che avevano le Province erano davvero importantissime e ancora lo sono, in parte: dalla viabilità alle strade, dall'edilizia scolastica alla formazione professionale, dall'ambiente alla gestione del territorio.

non abbiamo la possibilità di fare in modo che le Province possano dare risposte ai piccoli Comuni. Se penso alla mia Lombardia, ci sono Comuni che non possono avere un rapporto diretto con una Regione che ormai ha che ormai ha superato i 10 milioni di abitanti. La legge Delrio prevedeva un Presidente in carica per quattro anni e un consiglio provinciale in carica due anni,

altre vadano al voto per eleggere il Presidente e altre ancora per eleggere solo il consiglio provinciale: in questo modo si

ma sappiamo che quei servizi che le Province andranno ad amministrare (finché non verranno tolti) serviranno ai Comuni e ai nostri cittadini e allora una risposta va data immediatamente. Consapevole che

si faccia un'indagine conoscitiva, un approfondimento veloce, che renderà chiaro che se vogliamo aiutare i nostri amministratori che hanno un contatto diretto con i cittadini (sindaci e consiglieri comunali), dobbiamo dare anche a loro delle Province in grado di sostenere quel lavoro. Concludo dicendo che Forza Italia e anche altre forze politiche (la Lega in particolare) hanno presentato disegni di legge che vanno nella direzione dell'elezione diretta delle Province; si può fare con le elezioni europee senza costi per il Paese e quindi su questo chiedo davvero un salto di qualità. Abbiamo fatto una frittata e abbiamo creato un mostro che oggi è stato addirittura peggiorato nei suoi contenuti: facciamo in modo di rimediare, diamo dignità. Se qualcuno pensa che le Province siano inutili le cancelli, subito; se pensa che possano ancora servire - come pensiamo noi -

Le destinazioni balneari sono le preferite dal 68 per cento dei turisti, che si dichiarano molto soddisfatti dei servizi offerti, con ben 30.000 imprese e oltre 100.000 addetti nel settore. Evito i riferimenti normativi, perché non è la prima volta che parliamo della direttiva Bolkestein in Aula e ci vorrebbe molto più tempo di quello che ho a disposizione. Vorrei però nuovamente rimarcare alcuni punti fondamentali. Lungo tutta la nostra Penisola gli stabilimenti balneari rappresentano un comparto economico fondamentale, che non può essere lasciato in balia di una normativa ancora incerta, né tantomeno in attesa di tavoli o riunioni tecniche che ad oggi non è dato sapere quando avverranno. Occorre una legge di riforma che dia garanzia a queste imprese e che tuteli le specificità della loro attività. Nel corso degli ultimi decenni gli operatori balneari hanno migliorato, con il proprio lavoro, sacrifici e investimenti, l'aspetto e la funzionalità delle nostre coste, fino a renderle il simbolo dell'eccellenza turistica che tutto il mondo ci invidia. Questo patrimonio, che non è soltanto economico, ma culturale e direi addirittura identitario del nostro Paese, rischia di essere annientato, distrutto, perso per sempre. perciò nostro dovere evitare che ciò accada, tutelando le migliaia di piccole imprese, spesso a conduzione familiare, che hanno dato vita e corpo al settore. Infatti, non stiamo difendendo le *lobby*, i grandi fondi di investimento o i poteri forti, ma solo e soltanto le nostre famiglie italiane, che ormai da troppo tempo si trovano in una situazione di palese incertezza. Noi di Forza Italia, con in testa il presidente Silvio Berlusconi, siamo da sempre al fianco dei lavoratori e del mondo del lavoro. Purtroppo - e mi dispiace - non possiamo dire altrettanto di voi, che avete solo creato danno al mondo del lavoro, a partire dal cosiddetto decreto dignità, per proseguire con la confusione a riguardo delle graduatorie degli insegnanti (diplomati magistrali, TFA, sostegno eccetera), fino ad arrivare all'assurda

finestra"). Dichiaro chiusa la discussione generale. Come stabilito dalla Conferenza dei Capigruppo, la discussione del provvedimento riprenderà domani alle ore 9,30 con la replica del rappresentante del Governo.

Signor Presidente, colleghi senatori, da oltre vent'anni gli abitanti del Comune di Troia, in provincia di Foggia, e delle zone limitrofe a questo Comune convivono con una vera e propria bomba ecologica, che è costituita da una discarica abusiva sorta in località Giardinetto di Troia, nell'area dell'*ex* laterificio, una fabbrica di laterizi. In questo sito e, quindi, nei capannoni abbandonati e nei piazzali, sono stati stoccati e interrati in maniera illegale circa 300.000 tonnellate di rifiuti tossici, nocivi e pericolosi, provenienti praticamente da tutta Europa. I capannoni purtroppo sono aperti, perché ormai sono abbandonati da molti anni, e i rifiuti sono esposti alle intemperie, cosicché quando si verificano episodi meteorologici avversi di una certa intensità le cosiddette bombe d'acqua, l'ultima delle quali si è verificata a metà agosto scorso - sussiste il grave pericolo che le acque meteoriche e i venti portino questi rifiuti anche a notevole distanza dal sito, con ovvio e grave pregiudizio per la salute dei cittadini. Per quasi vent'anni questo problema, purtroppo, è stato praticamente ignorato, ma finalmente proprio in questi giorni in Regione Puglia si sta valutando il progetto presentato dal Comune di Troia per la caratterizzazione dei rifiuti presenti nel sito e per la bonifica dello stesso. I fondi a disposizione sono quelli del programma azione 6.2 Por Puglia FESR-FSE 2014-2020, Asse VI. Nei mesi scorsi un altro progetto presentato dal Comune di Troia, relativo agli interventi della tipologia A del bando, che prevedevano la messa in sicurezza di emergenza e misure di prevenzione di siti in presenza di sorgenti primarie e secondarie di contaminazione, purtroppo era stato bocciato. Oggi, invece, il Comune partecipa, unitamente ad altri Comuni esclusi, ad una prima fase della richiesta di fondi per la messa in sicurezza e noi auspichiamo ovviamente che il progetto questa volta sia meritevole di approvazione e che, conseguentemente, possa finalmente avere inizio questa importante opera di bonifica del territorio troiano. Questo per dare una risposta concreta a tutti i cittadini, a quelli che si sono battuti per tanti anni, per quasi vent'anni, in questa battaglia di giustizia e di legalità, ai comitati, agli attivisti del MoVimento 5 Stelle, ma soprattutto ai cittadini sfortunati che si sono ammalati in questi anni proprio a causa dei rifiuti presenti nella discarica abusiva. Concludo. Vigileremo affinché le attività, di caratterizzazione prima e di bonifica poi, siano svolte nel più breve tempo possibile e nella maniera migliore. Il nostro unico obiettivo è la salute dei cittadini. *(Applausi Signor Presidente, care colleghe, colleghi, nello Yemen da più di tre anni si sta combattendo una guerra tra una minoranza sciita *houthi* e il Governo Hadi, che rappresenta l'ala sunnita, quindi vicina all'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita è un Paese in cui prevale il wahabismo, che è la dottrina più radicale dell'Islam; una dottrina che i sauditi stanno tentando di estendere finanziando gruppi jihadisti e terroristi. Le vittime della guerra in Yemen sono almeno 10.000. I bambini stanno subendo pesantemente le conseguenze dirette e indirette di questa aggressione. Save the Children ha calcolato che ogni dieci minuti nello Yemen muore un bambino per fame e malattie causate dal blocco della coalizione saudita. Presidente, sono 50.000 i bambini malnutriti che quest'anno rischiano di perire e complessivamente sono più di 8 milioni i civili in grave pericolo a causa di mancanza di generi alimentari. Nel 2016 il Ministro della difesa del Governo Renzi era Pinotti; in quell'anno raddoppiarono le esportazioni italiane di armi. Infatti, nel 2015 l'Italia ha venduto all'estero armi per un valore pari a 7,9 miliardi di euro; nel 2016 il totale è stato di 14,6 miliardi, una vendita soprattutto verso quelle monarchie del Golfo che di certo non possono essere considerate un faro di democrazia, in particolare la citata Arabia Saudita, un Paese che ha prodotto personaggi come Bin Laden, ma anche 15 dei 19 dirottatori dell'attentato dell'11 settembre 2001. Eppure all'Arabia Saudita nel 2016 abbiamo venduto armi per 427,5 milioni di euro, tra cui 21.822 bombe prodotte in Sardegna; bombe che ogni giorno uccidono donne, bambini e uomini. Questa è una vergogna inaccettabile. Come ha ricordato il mio collega Lucidi, l'Arabia Saudita è un Paese accusato da ONU, Unione europea e Amnesty International di crimini di guerra in Yemen. Tale vendita di armi viola la legge n. 185 del 1990, che espressamente vieta di esportare armamenti verso Paesi in stato di conflitto. Sotto questo punto di vista, Luigi Di Maio e il ministro Trenta sono stati chiari: il cambiamento ci sarà anche in questo ambito. Concludo dicendo che noi non abbiamo più intenzione di continuare a sporcarci le mani di sangue e interverremo legislativamente per rafforzare tale divieto, nel rispetto dell'articolo 11 della Carta costituzionale.

ho chiesto di intervenire per portare a conoscenza dell'Assemblea l'esito del ricorso al Consiglio di Stato relativo al pronto soccorso di Città della Pieve. Riepilogo brevemente i fatti. Il 1° marzo 2017 la Regione Umbria, nell'ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera, decide la chiusura del pronto soccorso del Comune di Città della Pieve; un pronto soccorso che serve un'area di 12 Comuni, 60.000 abitanti, un'area disagiata, con difficoltà nelle vie di comunicazione e distante da altri presidi. Nel maggio del 2017 il sindaco del Comune di Montegabbione, Fabio Roncella, un Comune che è a 10 chilometri da Città della Pieve, ricorre al TAR,

Nel febbraio del 2018 il comitato e il Comune vincono il ricorso, perché il TAR stabilisce che il diritto costituzionale alla salute, il diritto ad aver difesa la vita da un pronto soccorso che possa permettere un intervento in tempi brevi, non può essere in alcun modo oggetto di tagli e riorganizzazioni sul piano amministrativo e solo con finalità di tipo economico e finanziario. nel febbraio del 2018, ma casualmente, verso la metà di marzo del 2018, la Regione dell'Umbria, invece che riconoscere i diritti dei propri cittadini, decide di ricorrere al Consiglio di Stato, ritenendo, come ha sostenuto l'assessore alla salute dell'Umbria, che le tabelle gli davano ragione e che erano più forti del diritto alla salute dei cittadini. Il 26 luglio c'è stata

è legale, ma non è giusto. Allora chiedo al Parlamento di prendere coscienza di questo, perché bisogna fare in modo che il diritto alla salute, sancito dall'articolo 32 non sia solo riconosciuto, ma sia effettivamente garantito, perché è dovere del Parlamento fare in modo che le scelte non siano semplicemente legali, ma che siano giuste e nell'interesse dei cittadini. È dunque importante che il Parlamento intervenga, perché fatti come questo - ci sono stati morti in quella zona

Presidente, colleghi senatori, voglio raccontare del signor Mario Lister, cittadino gradese di settantadue anni, perché mi sento in dovere di approfondire un drammatico evento, sepolto tra le righe del tempo. Era il 18 dicembre 1998, quando il fratello Giuseppe, detto Pino, e un collega di Lodi alla guida di una *jeep* nei pressi di Brazzaville, in Congo, sono stati coinvolti in una rivolta ancora oggi non attribuibile. Dai rapporti sembrerebbe che il lodigiano sia stato ucciso sul colpo da arma da fuoco, mentre si dice che Pino, ferito, sia stato trascinato via dagli aggressori e da quel momento è sparito per sempre. Pino era geometra e si trovava a Brazzaville per motivi di lavoro, nel settore edile. I carabinieri della stazione di Grado, in provincia di Gorizia, dissero allora che la Farnesina aveva motivo di ritenere che Giuseppe Lister fosse rimasto vittima di un'imboscata da parte dei ribelli congolesi e che era sparito senza lasciare traccia. Riferirono però di aver trovato la fotocopia della sua patente sul ciglio della strada dove era venuta l'aggressione. Nel corso del tempo sono state presentate due interrogazioni parlamentari e nel frattempo Mario, il fratello, ha speso ben 8 milioni delle vecchie lire per chiamare tutti i numeri telefonici pertinenti al caso, dalla Farnesina all'ambasciata italiana in Congo; ha contattato anche il Vaticano, ma mai nessuno è stato nemmeno in grado di dire se Pino, ovvero Giuseppe Lister, fosse vivo o morto. La risposta era sempre la stessa, come un vecchio disco rigato: "Se ci saranno novità, la chiameremo noi". Giuseppe, allora, conviveva con una signora congolese dalla quale sembrerebbe che abbia avuto un figlio, attualmente residente a Piacenza. Eppure nemmeno il ragazzo, né la madre hanno fornito una risposta sulla scomparsa di Pino. Il caso Lister arriva anche al Parlamento europeo che chiede l'intervento del ministro congolese Cécile Kyenge, ma la signora Kyenge non ha nemmeno mai risposto. Morte presunta. Osservo questa povera anima rassegnata, seduta davanti a me, che ancora una volta ha deciso di raccontare il suo dolore a una perfetta sconosciuta, nella speranza di poter chiudere un lutto mai conclamato. Attualmente, la sorte di Mario è simile al destino dei familiari dei caduti che si inchinano solennemente davanti al Monumento del Milite Ignoto, baciando il marmo freddo per sentire l'illusorio tepore di una finta ed impossibile rassegnazione che non può scaldare né recare pace all'anima. Ma le vittime del lavoro all'estero non hanno monumenti, né medaglie. Per loro solo la profonda ferita tatuata sul cuore